ordine del giorno: Seguito della discussione dei disegni di legge: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche (1611) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, alcuni emendamenti ed i relativi subemendamenti. Questa mattina gli ulteriori emendamenti presentati dal relatore sono stati trasmessi ai Gruppi. Il termine per la presentazione dei subemendamenti, inizialmente fissato da questa Presidenza per le ore 18 di oggi, su richiesta dell’opposizione, accettata dalla Presidenza, viene prorogato fino alle ore 21 di questa sera. Non appena scaduto tale termine, la Presidenza rinvieraalla Commissione giustizia i predetti emendamenti e relativi subemendamenti, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento. La Commissione giustizia e autorizzata a convocarsi, sin dalle ore 8 di domani, per pronunziarsi sugli emendamenti medesimi e relativi subemendamenti. E[` ]ugualmente autorizzata a convocarsi la 5ª Commissione permanente per l’espressione del parere sugli emendamenti. La seduta antimeridiana di domani non avraluogo. L’Assemblea tornera a riunirsi domani pomeriggio, alle ore 15, per il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo e del lavoro posto in essere dalla Commissione.

di questa seduta non avranno luogo interventi in discussione generale, che riprendera domani alle ore 15.

e non marginalmente, anzi direi sostanzialmente – il testo che sara poi all’esame dell’Aula. E[]questa la ragione per la quale noi riteniamo non opportuno svolgere una discussione

conoscendo anche il suo scrupolo nell’applicazione del Regolamento e la sua attenzione circa il fatto che si creino precedenti che possano essere impugnati anche nel tempo a seguire e che noi possiamo considerare non corretti, mi permetto di dirle che, per un’esigenza probabilmente di natura puramente sostanzialistica, estata autorizzata, nella seduta del 31 maggio, la presentazione di subemendamenti – ovviamente sotto il profilo sostanzialistico l’opposizione non ha sollevato la questione in Aula – ad emendamenti che non erano di origine ne´

ho ritenuto di doverne parlare qui, in Aula, per evitare che su questa si crei un precedente al quale l’attivita` successiva del Senato potrebbe essere legata.